Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare la Conferenza dei Capigruppo per aver iscritto all'ordine del giorno questa mozione relativo tema, certamente non esaustiva per il contenuto ma utile per aprire una discussione proficua con il Governo. Sono passati poco più di trenta giorni dal 24 agosto 2016, quando un sisma di magnitudo 6.0 ha colpito una vasta porzione dell'Appennino centrale tra le Province di Rieti, Ascoli Piceno e Perugia e ha coinvolto alcune decine di Comuni collocati nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo provocando i danni più ingenti nei Comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Il Sistema nazionale di protezione civile ha risposto ancora una volta con efficienza ed efficacia già dai primissimi momenti successivi al sisma, dimostrandosi fiore all'occhiello del nostro Paese e a esso va il nostro più sentito ringraziamento. In questo momento il lavoro della Protezione civile e del commissario governativo alla ricostruzione Vasco Errani sta procedendo congiuntamente, legando le risposte all'emergenza al percorso della ricostruzione per consentire un pronto ritorno alla normalità per cittadini e imprese, e l'avvio della prima fase delle sistemazioni abitative temporanee. Noi crediamo che il Governo abbia operato e stia operando bene e che serva oggi orientare la procedura di ricostruzione dei territori colpiti attorno a cinque imperativi chiave: qualità massima ed efficienza degli interventi, con il massimo rispetto possibile dell'identità dei luoghi e degli edifici; democrazia, attraverso una responsabilizzazione delle comunità locali e di tutti i livelli istituzionali presenti, facendo affidamento sulla responsabilità degli eletti; trasparenza, per mezzo di piattaforme informatiche per la gestione di tutte le risorse e la rendicontazione puntuale degli interventi; legalità, attraverso la creazione di meccanismi di selezione e controllo delle imprese incaricate dei lavori; equità, ovvero corresponsione del dovuto ai cittadini e alle imprese di tutte le comunità colpite. In questa direzione va apprezzato il lavoro di ascolto sul cosiddetto progetto Casa Italia, così come la scelta del coordinamento affidata al professor Giovanni Azzone, rettore del Politecnico di Milano, con il supporto di altre competenze ed esperienze. Noi crediamo che il progetto debba partire, però, da una verifica seria delle esperienze passate che, pur tra mille difficoltà ed errori, il nostro Paese ha saputo realizzare, con l'obiettivo di definire non tanto dei modelli, quelle correzioni di metodo e contenuto che consentano di varare e realizzare un piano dai risultati importanti e certi. Il Gruppo del Partito Democratico ha inteso portare all'attenzione dell'Aula e del Governo alcuni punti politici di indirizzo che reputa prioritari, e che si augura possano essere condivisi anche dagli altri Gruppi. In primo luogo, il perfezionamento ulteriore del Sistema nazionale di protezione civile, attraverso il sostegno a una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge delega, attualmente all'esame delle Commissioni la e 13a del Senato, al fine di migliorare un sistema che già rappresenta un'eccellenza italiana, ma che ha bisogno di importanti semplificazioni, completando la definizione dei ruoli e delle competenze delle Regioni, degli enti locali, del volontariato e della cittadinanza. In secondo luogo, abbiamo bisogno di rendere maggiormente efficaci le norme di carattere preventivo finalizzate al miglioramento sismico degli edifici, contenute già in diversi provvedimenti emanati nel corso anche degli ultimi anni, come - ad esempio - le norme per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, che questo Governo ha voluto sostenere in modo concreto. La cifra di 963 milioni di euro, anche se cospicua rispetto al passato, rappresenta una minima percentuale del fabbisogno necessario per il completo adeguamento sismico degli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture strategiche. Penso anche alle opportunità offerte dalle norme di carattere fiscale, come l'ecobonus. E proprio su questo provvedimento, in questa Aula, qualche mese fa si è discusso della sua efficacia e il Governo si è impegnato a darvi continuità per tre anni per sostenere così le ristrutturazioni e le riqualificazioni energetiche anche dei condomini. A nostro avviso, si potrebbero cambiare e semplificare i criteri e i meccanismi vigenti, estendendo le incentivazioni al 65 per cento anche agli adeguamenti e consolidamenti sismici, prevedendo norme specifiche per i soggetti incapienti. In terzo luogo, chiediamo al Governo di pianificare il fabbisogno pluriennale di risorse pubbliche e private, per dare seguito e continuità nel tempo alle proposte inserite nel progetto Casa Italia, indicando da subito le misure stralcio da prevedere negli strumenti finanziari già in discussione per il 2017. Si è parlato di sisma-bonus, ma non ci interessa una disputa nominale quanto la sostanza degli atti. Pensiamo che si possa considerare l'estensione del meccanismo ipotizzato da ENEA per gli interventi di efficientamento energetico dei condomini anche alla messa in sicurezza antisismica. Noi pensiamo che serva Noi pensiamo che serva infine sostenere il piano nazionale di prevenzione antisismica individuato nel 2009, con altre scelte strategiche che riguardano l'adozione del fascicolo di fabbricato e la certificazione sismica obbligatoria. Come Partito Democratico, a prima firma del collega Filippi, abbiamo presentato sul tema due specifici disegni di legge: uno contenente disposizioni per la riduzione della vulnerabilità sismica dei centri storici; l'altro per l'adeguamento sismico degli edifici privati ad uso residenziale e, quindi, l'istituzione del fascicolo di fabbricato. Si tratta di proposte concrete, frutto del contributo di tante competenze che mettiamo a disposizione del Parlamento e del Governo per dare gambe solide ad alcune delle scelte future delle scelte future del progetto Casa Italia: un progetto che si candida a diventare ambizioso, lungimirante e strategico per la sicurezza del nostro Paese. Investire risorse in prevenzione, anche quella non strutturale, anziché nella riparazione dei danni, significa investire sul futuro dei cittadini e delle imprese di questo Paese. È una sfida che possiamo vincere tutti assieme unendo le migliori competenze, intelligenze ed esperienze italiane al servizio di una buona causa comune.

è arrivato il momento, superata la prima fase di emergenza *post* terremoto e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite, di affrontare la delicatissima e lunga fase della ricostruzione. Bisogna garantire la celerità e la correttezza dell'opera di ricostruzione e il Governo deve dare subito certezze sul piano normativo.

le garanzie sulle risorse che saranno messe a disposizione nei prossimi anni. È indispensabile scongiurare il rischio grave di una ricostruzione poco trasparente e gestita dal Governo in modo autonomo ed eccessivamente centralizzato. È necessario garantire, infatti, la costante e piena partecipazione, nonché il consenso degli enti territoriali e delle comunità locali nelle scelte della ricostruzione e dell'eventuale trasformazione urbana. Pesa ancora su di noi e su quelle popolazioni l'esperienza dell'Aquila. Circa la modalità di ricostruzione, è necessario favorire la ricostruzione del patrimonio perduto, nelle condizioni originarie per tipologie e uso dei materiali, e comunque in coerenza con l'architettura tradizionale, salvaguardando certamente gli edifici di pregio storico e artistico, ma anche i complessi e i singoli edifici e manufatti non solo di antica formazione, anche se non di particolare pregio architettonico, ma rappresentativi della storia e della cultura delle comunità agricole. Bisognerà quindi affrontare una serie di nodi - lo dico subito - compreso il fatto che proprio nei borghi, nei centri storici di Amatrice,

perché, pur garantendo il rispetto della trasparenza e della concorrenza, occorre individuare specifiche misure a sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione locali, il più possibile coinvolgendole nella ricostruzione del territorio. tocca a noi oggi affrontare finalmente la questione della prevenzione. I frequenti eventi calamitosi che colpiscono il nostro Paese mettono in luce la drammaticità della fragilità del nostro territorio e la necessità di una ormai improcrastinabile messa in sicurezza complessiva degli edifici e del territorio stesso. Questa per noi è la vera, grande opera pubblica di cui ha bisogno il Paese. E lo dico con forza nel momento in cui si rilanciano opere assurde come il ponte sullo Stretto: la priorità assoluta per questo Paese è la tutela del suo territorio e la messa in sicurezza degli edifici per salvare le vite e la bellezza dell'Italia. L'Italia è uno dei Paesi a più elevato rischio sismico sia in Europa che a livello mondiale, e questo dipende non soltanto dalla frequenza e dall'intensità dei terremoti, ma anche dalla elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio. manca nel nostro Paese la cultura della prevenzione, che consentirebbe di limitare gli effetti drammatici degli eventi naturali.

Questi sono i dati che ci dicono che non dovremmo avere dubbi e che bisognerebbe presentare subito un piano decennale per la messa in sicurezza del territorio, che permetterebbe un investimento certo e sicuro. Desidero ricordare che, solo nel triennio 2010-2012, sono stati spesi più di 3,5 miliardi di euro all'anno per i terremoti.

Bisognerebbe dunque garantire la piena detraibilità del 65 per cento delle spese per l'adeguamento sismico dei condomini; assumere finalmente iniziative per prevedere l'istituzione obbligatoria del fascicolo del fabbricato

Bisognerebbe dunque articolare un insieme di interventi, con un combinato disposto di investimenti pubblici e agevolazioni fiscali,

assolutamente possibile - e un Paese serio non può che fare questo - articolare un piano. È stato presentato un immaginifico progetto, denominato Casa Italia. Speriamo davvero - non lo diciamo per partito preso - che non sia

gravissimi problemi per le aziende, soprattutto quelle agro-zootecniche, che solo nella zona di Amatrice sono più di 600. Ci sono danni agli edifici aziendali, e i danni alla viabilità creano ulteriori danni.

commissario straordinario, nonostante le gravissime criticità sollevate per la gestione del terremoto dell'Emilia-Romagna. che prorogherà per tre anni - bontà sua, dopo gli anni che noi lo andiamo ripetendo - l'ecobonus anche per quanto riguarda l'adeguamento antisismico degli edifici. Ha poi annunciato un non meglio precisato progetto casa per il futuro. È necessario prendere provvedimenti chiari e urgenti immediatamente, da un lato, per il caso specifico, e quindi per portare ristoro a quei territori; predisponendo un protocollo unico nazionale di intervento in modo che non si intervenga ogni volta caso per caso. Bisogna prevedere un fondo di rotazione nella prossima legge di stabilità, al fine di supportare anche gli interventi minori per la riparazione, ripristino e la ricostruzione degli immobili. Bisogna adottare iniziative per concedere indennizzi alle attività produttive danneggiate. Benché l'Europa li abbia valutati come aiuti di Stato, dobbiamo trovare il modo per poter aiutare anche le aziende a riprendersi e a rientrare dal danno che hanno subito. Bisogna attivarsi per creare una zona franca urbana in quelle aree; promuovere strumenti di partecipazione alla ricostruzione, ed essere certi che chi collaborerà alla ricostruzione

il quadro è chiarissimo. Abbiamo dei dati estremamente allarmanti. L'ingegnere sismico Alessandro Martelli ha valutato che l'80 per cento degli edifici in Italia non è idoneo. È stato valutato che una scuola su tre ricade in aree ad alto e medio rischio sismico, ma che solo l'8 per cento è

per le costruzioni in zone sismiche, una classificazione antisismica agli edifici e, soprattutto, quantificare le risorse necessarie all'adeguamento antisismico. Non abbiamo attuato questo piano; non abbiamo messo mano a questo importantissimo lavoro. Ci manca la base, perché dobbiamo aggiornare la carta delle sismicità di tutto il territorio e avere una mappatura certa degli edifici

dare una valutazione, come avviene per la classe energetica, in merito alla classe antisismica edificio per edificio. Un ingegnere, di cui adesso purtroppo non ricordo il nome, ha affermato che sarebbe necessario che, vicino alla targhetta del civico delle strade,

più fare degli *spot* che hanno termine annuale o triennale.

nelle transazioni immobiliari e per tutte le richieste di autorizzazioni edilizie. Infatti io devo sapere dove sto mettendo mano e quale sia la classificazione antisismica di quell'edificio prima di fare eventuali aumenti volumetrici (che adesso si potranno fare una con CILA), il che è gravissimo, perché non si saprà dove si sta agendo. Bisogna inoltre predisporre gli opportuni strumenti legislativi volti ad inibire la cessione di immobili sprovvisti di fascicolo del fabbricato e bisogna quindi informatizzare tramite il SIT, il il sistema informativo territoriale a livello nazionale, la mappa degli edifici che si trovano in zone sismiche e a rischio idrogeologico.

Signor Presidente, illustri colleghi, rappresentanti del Governo, il dibattito odierno verte su una questione assolutamente seria seria che non necessita di retorica, di populismo o di demagogia. È una questione sulla quale il Parlamento oggi dovrà esprimersi e dovrà farlo, a mio avviso, nella maniera più unitaria possibile per dare un contributo serio, attraverso un atto di indirizzo che costituisca per il Governo una sorta di programma di lavoro.

relative agli immobili ma anche al nostro territorio. È un programma ambizioso, il cui costo è valutato in circa 100 miliardi di investimenti e che necessita sicuramente di diversi decenni per essere espletato.

che vanno verso una semplificazione delle procedure di ricostruzione delle aree terremotate ad Amatrice e negli altri paesi interessati sì che definiscano, in assoluta sintonia con le comunità locali, non soltanto - per l'appunto - le procedure ma soprattutto le modalità. Siamo dell'idea che si debba ricostruire com'era e dov'era, certamente rispettando l'ambiente, la qualità e l'identità architettonica preesistente, tutelando il paesaggio, cercando, in una parola sola, di non far disperdere la memoria di quelle popolazioni.

Questo terremoto, di fatto, serve a cambiare un approccio che la politica ha sempre avuto nei confronti di queste calamità, superando il tabù della differenziazione tra prime e seconde case. Abbiamo Abbiamo il dovere di dare una risposta in tempi certi, ma abbiamo anche il dovere di evitare quanto - ahimè - accaduto precedentemente nel nostro Paese. Mi riferisco alle ruberie, alla corruzione, all'attenzione delle mafie che, in casi di questo genere, come torme di sciacalli si avventano alla ricerca di un facile guadagno e di un facile bottino.

chiaramente, ognuno di noi deve fare il proprio dovere. Il dovere della politica è l'assunzione di responsabilità, senza se, senza ma e senza paure. Il dovere della magistratura

anche se, personalmente, appartengo a coloro i quali ritengono che l'Autorità anticorruzione non possa e non debba essere evocata a ogni piè sospinto, ma debba rappresentare una risposta a situazioni emergenziali, una risposta, magari preventiva, nell'individuare modalità che incoraggino la trasparenza e che tutelino la legalità, ma che non possa e non debba mai sostituirsi alla primazia della politica. Abbiamo il dovere, signor Presidente, di evitare quanto accaduto in vaste aree del Paese in esperienze precedenti. che le aree terremotate diventino luoghi di sperimentazione e, magari, un luogo di architetture libere, nei confronti delle quali non ho assolutamente nulla in contrario ma che, in aree del Paese e in esperienze precedenti, hanno creato delle vere discrasie con il linguaggio dei territori e, quindi, le coscienze dei cittadini terremotati. Cittadini terremotati che, in taluni casi, sono stati terremotati due volte: disastrati per la calamità naturale e disastrati per l'intervento operato dallo Stato in materia assolutamente disastroso. Nella nostra mozione abbiamo individuato i mezzi tecnici. Sono convinto che la legge di stabilità rappresenti una occasione importante. Dobbiamo procedere alacremente alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, degli edifici privati, del nostro patrimonio storico artistico e culturale. dobbiamo procedere in tempi celeri. Certo è che il Paese non può più aspettare i ritardi della politica e, soprattutto, la distrazione dello Stato. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Pelino per illustrare la mozione n. 632. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci troviamo riuniti questa mattina a parlare di un argomento che tocca la sensibilità di tutti noi: il tragico sisma che ha colpito il Centro Italia durante una notte che si preannunciava come una tipica preannunciava come una tipica e serena notte d'estate e che invece si è trasformata in un incubo per migliaia di persone. Le conseguenze sono state davvero pesanti: sono stati rasi al suolo interi Comuni e frazioni limitrofe: Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Montegallo, Montemonaco, Montefortino e Amandola sono i Comuni più colpiti in termini di perdite di vite umane e risultano quelli che hanno subito i più gravi danni a edifici pubblici, storici e privati. Abbiamo avuto modo di commemorare, i primi di settembre, qui in quest'Aula, la perdita dei quasi 300 nostri italiani che in quella brutta notte hanno trovato la morte e non è mai troppo tardi per rivolgere ancora un pensiero a tutte le famiglie che piangono la scomparsa dei propri cari. Oltre alla vicinanza e alla solidarietà che noi possiamo esprimere, sappiamo bene di essere i rappresentanti delle istituzioni e questo non ci esime dal dover svolgere il nostro compito fondamentale, ovvero quello di vigilare sul piano che il Governo intende mettere in atto per la ricostruzione di tutti i territori territori che, in un colpo solo, si sono trasformati in tristi accumuli di macerie. Noi di Forza Italia esprimiamo apprezzamento per come il Governo ha gestito la fase dell'emergenza, grazie anche allo straordinario lavoro dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino, della Protezione

ai 3.000 cittadini sfollati che hanno trovato rifugio nei campi, nelle strutture allestite o presso gli alberghi. Ho seguito da vicino questa triste vicenda, però spesso mi sono imbattuta in commenti che inducono in errore. È noto che quando si verifica un fatto simile ad un altro si ha la tendenza a fare dei paragoni. Devo ammettere che trovo questa operazione alquanto semplicistica e fuori luogo. Si sente parlare del parallelismo tra quest'ultima catastrofe naturale e quella che ha colpito il mio Abruzzo nell'aprile del 2009, oppure con quella che ha interessato l'Emilia-Romagna nel maggio del 2012. Si tratta di un esercizio puramente teorico, perché la realtà, a mio modesto parere, è che ogni fatto ha delle caratteristiche precipue che lo distinguono dagli altri. Tanto è vero che un semplice elemento spiega bene l'inadeguatezza del descrivere le diverse situazioni attraverso i fiumi di inchiostro e di parole, ricorrendo ai raffronti comparativi. Il terremoto che ha colpito l'Abruzzo, e l'Aquila in particolare, ha causato circa 60.000 sfollati, una cifra oltremodo superiore rispetto ai 3.000 del terremoto di quest'estate. Non solo, ma anche la diversa configurazione territoriale rappresenta un elemento che non facilita la comparazione. Che siano 60.000 o 3.000, il nostro dovere, in primo luogo del Governo, è quello di predisporre un piano destinato alla ricostruzione, che venga esteso, oltre alla riedificazione e al ripristino delle abitazioni, al tessuto imprenditoriale, che rappresenta il primo motore da riaccendere per far ripartire l'economia dei territori colpiti. Occorre dunque che il Governo si impegni ad un costante monitoraggio di ogni fase della ricostruzione e ad un controllo continuo e meticoloso durante l'esecuzione dei lavori, soprattutto per evitare che ci siano infiltrazioni da parte della criminalità organizzata e, altresì, per scongiurare che le risorse pubbliche vengano sprecate; inoltre, ciò che viene ricostruito o ristrutturato dovrà essere assolutamente sicuro. A nostro avviso non c'è tempo da perdere. Chiediamo, infatti, al Governo e al presidente Renzi - che saluto in questo momento - di stanziare, già dalla prossima sessione di bilancio, le risorse adeguate per avviare e garantire la ricostruzione. Si stimano 4 miliardi di euro di danni ed è necessario dunque cominciare fin da subito. Quanto ai nostri cittadini, noi di Forza Italia chiediamo che si faccia il possibile per favorire, in tempi brevi, il rientro alla normalità della loro vita quotidiana. Per ottenere questo risultato occorre che il Governo, oltre ad aver deciso per la sospensione dei versamenti delle imposte e degli adempimenti tributari per tutti i contribuenti (persone fisiche, imprenditori, persone giuridiche), assuma l'impegno di estendere l'ombrello fiscale a diverse altre fattispecie, che non sono state affatto prese in considerazione nel decreto del Ministro dell'economia. Per esempio, tra gli altri, la sospensione del pagamento dell'IVA per tutti gli interventi volti alla ricostruzione e la sospensione del versamento dei contributi INPS e INAIL. In conclusione, va dato atto al Governo che la fase dell'emergenza è stata gestita in maniera adeguata. Va però detto che la fase della ricostruzione è quella più delicata, La mozione presentata dal Gruppo di Forza Italia intende dare un contributo all'individuazione delle priorità da affrontare e delle modalità per farlo.

il terremoto del 24 agosto 2016 che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ha avuto effetti devastanti,

ripetere, descrivono nella loro oggettività le dimensioni del dramma del 24 agosto scorso. Nei giorni successivi alla tragedia il Governo ha annunciato una serie di misure, alcune delle quali già abbozzate nella legge di bilancio per il 2017 come la proroga degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico, altre che confluiranno nel piano "Casa Italia", in modo articolato con interventi

che impegnava il Governo a dare stabilità, per il triennio 2017-2019, all'agevolazione fiscale del 65 per cento prevista per la riqualificazione energetica degli edifici. Il tema della prevenzione sismica in Italia è il punto nevralgico su cui anche il miglior piano di protezione civile e di pronto intervento deve confrontarsi, visto che in Italia il 70 per cento dei fabbricati è stato

a quello di Amatrice - con 4.900 vittime e circa 692.000 sfollati. Alla luce della letteratura disponibile sul rischio sismico e considerate le numerose esperienze del passato, ogni piano di prevenzione a lungo termine va attentamente meditato per non incorrere nel rischio che, tra il verificarsi delle catastrofi naturali e gli interventi di ricostruzione, siano posti in essere azioni o programmi di intervento che annientino l'economia locale delle zone colpite, desertificando i relativi contesti sociali. Penso che questa sia una preoccupazione del Governo, così come di tutte le forze politiche. Nel delineare interventi di mappatura delle zone maggiormente a rischio su cui intervenire prima di altre con piani complessi e articolati, si deve dunque procedere con estrema cautela, consapevoli dei lunghi tempi necessari per realizzare gli interventi annunciati, che poi si attuano magari dopo un decennio, con l'inevitabile crollo del valore degli immobili e la riduzione degli investimenti industriali e delle attività turistiche e produttive in generale. Il primo obiettivo da realizzare è quindi quello di non abbandonare il territorio, ovvero di non privilegiare una tipologia di interventi prima di un'altra. È necessario in modo organico le fasi della ricostruzione delle prime abitazioni, delle seconde case (che pure nel caso dei Comuni colpiti di recente sono importanti, perché mantengono un legame tra chi magari è venuto a vivere a Roma e cerca di ritornare nei propri luoghi di nascita), delle strutture produttive (comprese quelle turistico-ricettive) e delle infrastrutture pubbliche, in modo da non interrompere quei legami di cui dicevo prima. Occorre inoltre sottolineare che le recenti esperienze di catastrofi naturali che il nostro Paese ha vissuto, con particolare riferimento agli ultimi eventi sismici di Marche, Umbria e Abruzzo, vedono a distanza di anni i cittadini continuare a combattere con la malaburocrazia, cioè con una burocrazia lentissima, per accedere ai fondi per la ricostruzione. Nei casi peggiori addirittura le risorse destinate alle ricostruzioni sono terminate senza che i vari governi centrali e regionali avvicendatisi ne stanziassero di nuove. È ovvio - ma è bene ricordarlo e impegnare il Governo in tal senso

cento per l'efficientamento energetico, così come abbiamo cercato di fare anche con la mozione approvata a maggio dal Senato. Chiediamo inoltre di garantire misure speciali per la riqualificazione e l'adeguamento antisismico di tutti gli edifici pubblici, dando particolare priorità alle strutture sanitarie e scolastiche e, se necessario (sicuramente lo sarà), intervenendo presso la Commissione europea per reperire altre risorse.

che il Governo prevedesse misure per la prevenzione e il recupero del dissesto idrogeologico, più volte annunciate, ma mai realmente messe in atto. Chiediamo pure che il Governo possa garantire misure speciali per la ricognizione dell'effettivo completamento delle ricostruzioni dei danni causati dagli eventi calamitosi degli ultimi cinquant'anni, al fine di completare le opere avviate e le ricostruzioni degli edifici pubblici e privati tuttora non realizzate. chiediamo un impegno a prevedere una mappatura del territorio nazionale, in modo da conoscere l'ubicazione degli allettati gravi e dei disabili che in caso di emergenza non sono in grado di deambulare autonomamente, al fine di attivare specifiche forme di assistenza

Signor Presidente, la circostanza è particolarmente importante, grave e gravosa e ci deve sentire tutti partecipi in un accorato appello al Governo, quello di considerare

Considerare questa ripetizione nel tempo come la necessità di dare delle risposte preventive, in grado di evitare, com'è accaduto

stampa: abbiamo anche i fotografi in una postazione differente rispetto a quella usuale, perché evidentemente devono ritrarre anche qualche illustre senatore. E saluto per la sua presenza il senatore Renzo Piano, che per la seconda volta dall'inizio della legislatura ci ha raggiunto, con i fotografi a suo favore, che possano ovviamente suggellare questo sodalizio con il presidente Renzi. Presidente Grasso, ci aspettiamo dal Governo un'azione seria, perché il terremoto non ha solo colpito quelle famiglie, ma ha anche devastato un territorio, ha cambiato la vita di una generazione.

Ho trovato persone che, anche se colpite nuovamente dal terremoto, hanno espresso con grande fermezza la voglia di continuare a vivere in quelle terre, di non piegarsi rispetto ad eventi calamitosi che possono essere evitati,

Parallelamente, signor Presidente, occorre che vi siano azioni in grado di ricostituire il tessuto sociale e urbano che è andato perso con l'evento sismico. Non basterà ricostruire le case Non basterà ricostruire le case con i soldi; non basterà perché le persone che ci vivono dentro sono l'essenza di quei paesi. Non sono solo belle costruzioni, ma sono paesi fatti da belle persone, che si impegnano eroicamente a mantenere, in territori lontani dalle grandi città città che altrimenti sarebbero persi e condannati al declino, una storia, una tradizione, un modo di vivere, di cui andiamo fieri quando facciamo propaganda del *made* *in* *Italy* all'estero, ma di cui dobbiamo essere altrettanto consapevoli in questa circostanza. dare ora supporto a quelle popolazioni è un dovere per tutti i cittadini e la fiscalità generale deve impegnarsi seriamente, non solo alla ricostruzione ma anche per consentire che sia ricostituito il tessuto socioeconomico. Ci sono condizioni notevolmente differenti, a seconda di dove si esaminano gli effetti del terremoto, anche con dei paradossi. Se si attraversa l'Appennino ci si troverà

dietro i Monti Sibillini (penso a Norcia e alla Valnerina), ci si trova con case ancora in piedi, seppur con gente altrettanto devastata dal punto di vista della progressione economica o della possibilità di garantire

dobbiamo considerarli. Ho potuto vedere persone prendere già autonomamente sulle proprie spalle la responsabilità di pensare alla ricostruzione, senza attendere che arrivi lo Stato per ricostruire, ma - come dicevo prima - con grande dignità, cercando solo di avere regole facili tramite le quali poter dare ai propri figli una continuità in quei territori. Sono territori caratterizzati da un'economia rurale, umile e semplice,

possa esservi una nuova generazione di abitanti che resti lì. Non nascondiamoci che esiste anche una narrazione televisiva molto lontana dalla realtà.

sulla costiera adriatica, ma esistono anche coloro che vogliono restare e continuano a rimanere, a mille metri di quota e con l'inverno alle porte, perché non vogliono abbandonare i loro allevamenti

Ci siamo premurati di andare a parlare con i cittadini di queste zone, di raccogliere le loro richieste e le loro aspettative che consegniamo al Governo Non traditele solo per una fotografia o per un *selfie* sul giornale. Presidente Renzi, non traditele solo per avere un consenso da giornale: sarebbe una doppia morte per coloro che hanno perso la vita.

credo che nell'affrontare questa discussione dobbiamo partire da un dato di fatto, vale a dire che quello italiano è un ritardo epocale sul fronte della prevenzione antisismica e non perché non si sia speso per le ricostruzioni. Si calcola infatti che dal 1968 al 2012 si siano spesi 121 miliardi di euro, ma sono stati spesi con una logica emergenziale, mentre un piano antisismico che coinvolgesse edifici pubblici e privati e le stesse opere infrastrutturali strategiche sarebbe costato 100 miliardi di euro e quindi avrebbe fatto risparmiare soldi pubblici e soprattutto avrebbe salvato vite umane. Anche lo strumento messo in campo dal governo Berlusconi nel 2009, dopo il terribile terremoto dell'Aquila, si è dimostrato insufficiente: il fondo per la prevenzione dal 2010 al 2016 ha stanziato 965 milioni di euro, che secondo un rapporto della Protezione civile sono stati del tutto insufficienti, non coprendo nemmeno l'1 per cento del fabbisogno che sarebbe necessario per il completo adeguamento antisismico di tutte le costruzioni. Le linee guida del Governo dopo il terremoto del Centro Italia di agosto sembrano abbastanza delineate: ricostruzione nel rispetto delle identità dei luoghi, coinvolgendo le comunità, ma soprattutto senza deroghe al codice degli appalti e solo con imprese iscritte nelle liste di merito dell'ANAC, *open data* per monitorare gli interventi e l'uso dei 15 milioni di euro raccolti con le donazioni, politiche di sostegno alle imprese e programmazione urbanistica. Sono linee guida che il Governo intende seguire per la ricostruzione e sono linee sinceramente condivisibili per uscire dalla logica emergenziale con cui nei decenni passati sono stati affrontati

ovunque siano avvenuti, quindi non ci si limiterà ad indennizzare i danni verificatisi nel cratere del sisma, ma anche quelli che il terremoto ha provocato più lontano Entro l'anno dovrebbero poi arrivare le linee guida sulla classificazione sismica degli edifici ed è bene che non si vada oltre nei tempi perché di tempo, come ho già detto, se ne è perso anche troppo, non dopo questo terremoto, ma con i ritardi accumulati tanti decenni in cui si sono spese somme importanti senza mai varare un grande piano di consolidamento antisismico. Il commissario per la ricostruzione Errani ha annunciato la volontà del Governo di creare un meccanismo virtuoso basato su incentivi fiscali rafforzati e semplificati per avere la massima adesione al programma di adeguamento antisismico anche da parte di banche ed enti pubblici. A beneficiare del sisma-*bonus* saranno anche le seconde case e i condomini, ma anche gli enti locali che dovranno mettere in sicurezza gli edifici pubblici, a partire ovviamente da quelli di interesse strategico, tra cui, in primo piano, Un punto che va affrontato è quello del fascicolo del fabbricato che da troppo tempo è rimasto lettera morta. È assolutamente necessario renderlo obbligatorio senza che questo passaggio burocratico incida troppo sui bilanci delle famiglie. La soluzione potrebbe essere quella di inserire la spesa per la compilazione del fascicolo del fabbricato nel *bonus* 50 per cento sulle ristrutturazioni. Con la nostra mozione abbiamo cercato di dare un contributo di proposte per arrivare nel medio per scongiurare nuove catastrofiche distruzioni e soprattutto nuove vittime.

fiscalmente, che copra, tra gli altri, anche i rischi derivati dalle calamità naturali. prevedendo, a fianco dell'indispensabile intervento pubblico, l'entrata in scena di soggetti terzi come le compagnie assicurative, sottoposte al coordinamento di un'autorità pubblica, le quali per tutelare i propri interessi sarebbero ovviamente invogliate a spingere gli assicurati a comportamenti responsabili, tesi a contenere gli effetti dei disastri della natura. altri punti che incidono sulla trasparenza degli appalti e sulla programmazione di interventi di lungo periodo; non è infatti possibile che l'Italia resti indietro a Paesi come la Turchia e il Cile che, pur disponendo di un patrimonio abitativo qualitativamente molto inferiore, hanno già avviato piani trentennali di demolizioni e ricostruzioni.

molto puntuale e riguarda un'emergenza nell'emergenza. Come abbiamo visto nell'esperienza del terremoto del 24 agosto, ma anche precedentemente, la presenza di molte persone con disabilità disabilità è un ulteriore emergenza nel dramma generale. Questo ordine del giorno chiede di poter modulare anche

pre-*referendum* da parte di un Presidente del Consiglio che ormai tra poco prometterà lo stipendio anche a mio figlio che ha un anno,

gli 8 miliardi di euro vengano spesi per la ricostruzione nelle aree terremotate e la sistemazione antisismica dei territori classificati come aree sismiche.

opportunità e per scelte, e purtroppo chi viene in quest'Aula a bere il tè non ha la sensibilità di chi sta vivendo quei drammi

bensì come senatore a vita e credo che sia l'unica cosa con cui possa essere utile in quest'Aula un senatore a vita.

È importante che questo progetto sia di lunga durata. Naturalmente capisco: c'è un dramma, una tragedia accaduta poche settimane fa.

è sicuro per definizione. Questa è la ragione per cui credo che questo progetto generazionale sia importante e, tutto sommato, è forse un mestiere adatto ad un senatore a vita, perché sarò qui finché

è diventata più precisa, più scientifica e più attenta, man mano che le diagnosi sono diventate più precise. Man mano che esse sono diventate più precise, la chirurgia è diventata meno invasiva e distruttiva.

La diagnostica degli edifici è un punto di partenza, perché questa diagnostica così precisa consente subito di passare ad una cantieristica leggera.

Vi assicuro che si possono fare delle chiavi, che rinforzano gli edifici, senza distruggerli e spaccare tutto. Non mi voglio dilungare, ma quelli che da tra di voi capiscono di tecnica, sanno di cosa voglio parlare. Benvenuti nel mondo della contemporaneità. Sul tema della casa, bisogna passare dal mondo leggermente medioevale in cui viviamo, ad un mondo che ci appartiene. Perché è dunque così importante questa diagnostica e perché è importante fare i cantieri leggeri? C'è una ragione umana, molto importante: in tal modo non si devono allontanare le persone dalle loro case. Questa è la verità ed è qui che entra in gioco l'elemento inventivo. Vedete - lo sapete meglio di me - c'è una connessione fortissima tra la casa e chi la abita, tra le mura e chi ci sta dentro. È un'unità inscindibile e non è immaginabile separarle. Non allontanare le persone dalla casa significa immediatamente avere la possibilità di abbassare i costi di intervento: costi fisici, economici ma anche quelli umani. Sto parlando di un progetto che deve durare due generazioni; mi auguro che cominci subito, naturalmente, deve cominciare, ma qualcuno deve pensare a questi tempi lunghi, perché sono quelli che ci mancano. In Italia siamo bravissimi nell'emergenza immediata. La Protezione civile è uno degli esempi migliori che abbiamo al mondo; siamo leggermente meno bravi sul lungo termine. Quindi, questa idea di fare qualcosa che si possa fare senza allontanare la gente dalle proprie case rende il progetto molto più fattibile, anche sul piano pratico, evidentemente, sul piano umano ed economico. Bene, nella sostanza cosa propongo? Lo propongo - ripeto - nell'ambito del mio ruolo così com'è, con un gruppo di lavoro che è accanto a me e che lavora in questo senso, senza bisogno di nulla, se non stare assieme ed essere utili al Paese. A questo punto propongo di fare dieci prototipi. Vedete, nel mio mestiere - lo so benissimo - bisogna fare dei prototipi; non basta parlare, non bisogna nemmeno scrivere, non basta. Bisogna fare esempi, costruire dei prototipi. So benissimo come si devono costruire i prototipi: sono degli esempi. Bisogna costruirli lungo l'arco dell'Appennino, la zona sismica, che viene dai Balcani in realtà; ci accompagna ai Balcani. Bisogna scegliere attentamente

fa. Occorre partire da queste due famiglie e poi naturalmente bisogna parlare di tecniche costruttive: la pietra, il laterizio, la struttura mista, il cemento. Sono state costruite cose spaventose in cemento

L'idea è di costruirli nei prossimi anni, non nei prossimi cinquant'anni, in tempi brevi. Abbiamo la competenza per poterlo fare.

so come si fa. Si può fare, ma ci vogliono due o tre cose. La prima ovviamente è un'organizzazione, che però è possibile. Il nostro non è un Paese in rovina. È un Paese che può disporre annualmente, su un tempo lungo, *budget*. Non voglio entrare nei dettagli - non è mio compito - ma stiamo parlando di un patrimonio di 10 milioni di case. Questo è l'ordine di grandezza. Qualcuno dirà che sono otto, nove, Stiamo parlando di tutto il patrimonio residenziale che sta sulla spina degli Appennini e non solo, naturalmente. Un patrimonio fatto di borghi molto spesso. Ebbene, Ebbene, questo patrimonio di 10 milioni di edifici può essere messo in sicurezza - la sicurezza, la certezza non esiste con il sisma, ma la salvaguardia sì ma la salvaguardia sì - con un costo che ovviamente è limitato grazie al fatto che ho spiegato poco prima. Non entro nel dettaglio di quanti soldi ci vogliono, ma sono soldi che possono essere trovati facilmente nei bilanci di ogni anno. Sono soldi che rientrano immediatamente in circolazione: è come dare ossigeno, perché sono microfinanziamenti, microimprese, microcantieri. C'è anche bisogno di una macroimpresa, diciamo così: c'è bisogno di una grande organizzazione, ma sono soldi che rientrano immediatamente. Questo è un terreno su cui mi trovo meno a mio agio,

Ecco, «rammendo» è una parola un po' troppo umile, però di questo si tratta. Si tratta di cominciare e non smettere più e di vergognarsi di dimenticare i drammi, che passano, escono dalla cronaca e si dimenticano.

ma non è fatale che non si reagisca. Si dice che la natura è cattiva; la natura non è cattiva, né buona; è completamente indifferente, è completamente indifferente, però ha fatto una bella cosa: ci ha dotati dell'intelligenza, che è una cosa naturale. L'intelligenza ci ha consentito da quando esistiamo di coprirci, costruire dighe, argini e case per proteggerci. Difendiamoci, allora. Bisogna abbandonare il terreno della fatalità. Bisogna smettere di parlare di fatalità. Questo credo che sia un elemento culturale molto importante. C'è quella che definirei una responsabilità collettiva. Dobbiamo tutti metterci in testa che questa è una verità. Non possiamo nasconderci. Ci sono persone che non vanno a fare le analisi mediche per paura di sentirsi dire che sono malate.

Sono forse un osservatore privilegiato, ma ho quasi l'impressione che in Italia ci si sia assuefatti alla bellezza del nostro Paese. C'è una sorta di assuefazione per cui non ce ne rendiamo più conto. Forse gli italiani non si rendono più conto di che patrimonio abbiamo.

È una bellezza che non appartiene a noi, ma al mondo: è patrimonio dell'umanità. Me lo sento dire molto spesso: "Non vi sembra di essere dei custodi leggermente disattenti di tanto patrimonio"?

Ci sentiamo colpevoli solo per il tempo in cui piangiamo i morti. C'è qualcosa di sbagliato. Non si può andare avanti così. Bisogna cambiare qualcosa. Siamo dei custodi di una bellezza straordinaria che ci viene invidiata e di cui possiamo andare fieri. Non possiamo vantarcene perché non l'abbiamo fatta noi, ma l'abbiamo ereditata

Rischiamo, se non stiamo attenti, di essere eredi indegni. Non lo siamo, ma potremmo diventarlo se non stiamo attenti. Per questo ci vuole un progetto di lunga durata.

di difenderlo e di non dimenticare nel tempo, io sento questa responsabilità. È un privilegio enorme, è un grande onore essere senatore a vita.

il senatore Margiotta.

So quindi di cosa si tratta quando si parla di terremoto. Proviamo a mettere alcuni punti in linea, in linea, uno dopo l'altro. In primo luogo, il dipartimento della Protezione civile in Italia funziona, ha funzionato benissimo anche questa volta. Mi ha fatto piacere, per esempio, ascoltare un tributo in tal senso anche da parte della senatrice Pelino, segno che quando si parla del bene dell'Italia si superano le barriere di opposizione e maggioranza. Anche in questo caso voglio rendere un tributo a tutti coloro i quali,

nei momenti di emergenza in modo assolutamente concreto. È un punto di eccellenza della macchina del nostro Paese.

Vogliamo occuparci in modo sistemico e organico di questi temi. Non a caso il PD ha presentato in queste ore due disegni di legge a prima firma Filippi e Vaccari,

sono andato a Tokyo e lì è difficile vedere un edificio che abbia più di trent'anni perché non sanno dove andarlo a trovare. L'Italia è l'Italia, con la sua complessità, con la sua specificità,

E molto bene ha fatto a investire immediatamente il senatore a vita Renzo Piano che, con la sua presenza illustra quest'Aula. È un fuoriclasse, che dà valore al percorso Così come ha fatto bene a investire il rettore del Politecnico di Milano. Così come è un fuoriclasse di altra natura, sul piano amministrativo, lo stesso Vasco Errani, al quale il Presidente ha voluto affidare il difficile compito. È una sfida, non solo per la politica, ma per l'ingegneria, l'arte, il genio degli italiani. Proviamo a fare di questa tragica occasione una opportunità. Mettiamo al lavoro i nostri giovani. Studiamo bene i materiali, le tecniche costruttive, le metodologie di recupero. È chiaro che questa nostra generazione ha soprattutto il compito di mantenere il patrimonio edilizio. questo viene prima (e lo ripeterò in conclusione) delle grandi opere, ma senza rinunciare alle grandi opere, se vogliamo essere un grande Paese, ambizioso e non pauperistico. Lo ha detto meglio di me Renzo Piano. Si parta da una analisi

documentazione cartacea e basta: ha senso se parte, come ha detto appunto Renzo Piano, dai sondaggi sui calcestruzzi, sui materiali, soprattutto dai sondaggi sulle fondazioni. La legge che vogliamo approvare deve dire tutto questo.

il calcestruzzo utilizzato negli anni Cinquanta sia meno sicuro delle murature utilizzate nei secoli scorsi. Infatti, anche nel recente avvenimento, come avete visto, è stato proprio un edificio in cemento armato a crollare per primo. Quindi, bisogna lavorare sulle periferie e anche sulla qualità dei materiali che vengono usati lì. È ovvio che il programma di recupero e di messa in sicurezza debba partire dalle scuole. Anche il tema più volte sollevato, ancora una volta in maniera demagogica, della trasparenza è molto serio. Perciò abbiamo approvato un codice degli appalti e lo misureremo su questi temi, con attenzione anche in ordine alle costruzioni private. Non siamo di quelli che non fanno le Olimpiadi perché hanno paura di non poter garantire la trasparenza: vogliamo fare le cose e vogliamo farle in trasparenza.

Confido molto nel risultato. Ringrazio il collega Vaccari, il presidente Zanda e il Governo per questa iniziativa giustissima. Dopo ogni terremoto sembriamo svegliarci

Siamo presi da una sorta di vergognoso fatalismo per cui allontaniamo da noi il pericolo, perché pensiamo che a noi non succeda mai, che succede solo agli altri, lontano da noi. E magari si preferisce il cornetto in tasca alla rigorosa consapevolezza. Ho apprezzato molto il presidente del Consiglio Renzi e tutto il Governo che, a poche ore dalla terribile scossa delle 3,36, ha affermato la necessità di un programma nuovo: Casa Italia, appunto. Mai più farsi trovare impreparati dal terremoto che arriva a tradimento, magari di notte alle ore 3,32 come all'Aquila o alle 3,36 come il 24 agosto. Ti pugnala alle spalle e butta giù quello che trova debole e incapace a resistergli. Il terremoto se ne frega delle rassicurazioni mediatiche, arriva e basta. Non è, però, il terremoto che uccide; ad uccidere sono

danneggiati nel 2009 e ora nuovamente colpiti. Straordinario lo sforzo dei volontari e degli enti locali, eccezionale la generosità degli italiani. Mi chiedo però per quale ragione tutta questa bellezza e grandezza non le facciamo agire prima, invece che dopo. In questi anni e con questo Governo qualcosa

sono chiare ed emblematiche di quello che in positivo potrebbe accadere nel nostro Paese. Servono più risorse per più generazioni e un piano che abbia il senso della continuità e della stabilità. investire nella messa in sicurezza dei borghi delle nostre aree interne, a cominciare da quelle ad alto rischio sismico, anche in base alle diagnosi - come veniva detto - alle mappe di zonizzazione e microzonazione sismica. Casa Italia deve diventare la risposta con contenuti e tempi certi. La battaglia per il fascicolo del fabbricato che faccio dal 2009 non fu allora recepita. Ora che anche all'Aquila e in Abruzzo stiamo finalmente ricostruendo i centri storici, grazie alle nuove norme ed alle nuove risorse decise da questa maggioranza, cominciamo a intravedere la nuova città, ma ci siamo arrivati dopo anni con errori e inesattezze: facciamone tesoro. Bisogna avere una legge quadro (io l'ho presentata per l'Abruzzo); ci sono ottimi strumenti legislativi proposti dai colleghi, molte delle previsioni sono state già calate nelle leggi di stabilità e nei decreti enti locali. Queste esperienze vanno prese per ricavarne il meglio. Diciamoci la verità, ci preoccupiamo del pavimento, del colore delle mura, del garage o degli infissi, ma non ci chiediamo se la nostra casa ha solide fondamenta,

di fondo che chiama in causa responsabilità politiche e anche quella di tutti noi individui. I punti della mozione sono quindi giusti ed importanti: conclusione necessaria dell'*iter* della legge di riordino; orientamento della ricostruzione sui cinque imperativi chiave anche utilizzando le buone prassi conseguite in altre esperienze, come all'Aquila e altrove, dove abbiamo conseguito finalmente normative molto più adeguate: pensiamo, ad esempio, all'istituzione di zone a economia speciale (ZES) nelle aree colpite dai terremoti e dalle calamità naturali; vi è poi la necessità di uscire dalla logica delle ordinanze contraddittorie per avere una legge organica: non è possibile che a ogni terremoto cambino i diritti vi faccio un esempio concreto. Il terremoto del 2009, oltre a colpire le periferie, ha interessato decine di centri storici e di borghi. Per ricostruirli rapidamente, bene e con maggiori *standard* di sicurezza, non si può distinguere tra prima e seconda casa. Ora giustamente tutti parlano di ricostruzione anche delle seconde case: io sono d'accordo e farò questa battaglia. Desidero però ricordare che nei borghi d'Abruzzo terremotati le seconde case non furono finanziate: gli emendamenti che andavano in tal senso furono respinti. Conseguenza di quel comportamento è stato il blocco della ricostruzione dei centri centri storici, dove ci si obbligava a formare degli aggregati, ma dentro quegli insiemi il differente regime tra prime e seconde case di fatto bloccava le progettazioni. Solo con questo Governo abbiamo superato quell'*handicap*. Perché arrivarci dopo cinque anni,

fronte a un'altra grave situazione, interveniamo con energia, facendo tesoro di tutte le nostre esperienze Signor Presidente, abbiamo ascoltato con interesse il collega Piano

a progettare e costruire qualcosa da consegnare alla società: questo è sicuramente un buon approccio. Mi permetto sommessamente di ricordare al collega Piano che abbiamo avuto illustri esempi

La diagnosi, che lei giustamente ritiene essere fondamentale per costruire questi prototipi e dare una risposta, in talune parti del Paese è stata fatta. Voglio citare la mia Regione - in questo caso come prototipo, visto che vogliamo parlare di prototipi - in cui il piano territoriale regionale è stato approvato insieme a tutti i piani piani conseguenti delle Province, che hanno individuato in maniera specifica quegli elementi che dovrebbero costituire l'intera pianificazione del territorio e, di conseguenza,

siamo contenti che finalmente in quest'Assemblea ci sia un dibattito che, seppur in parte un po' da sognatori,

che ciò che stamattina ci è stato rappresentato dall'architetto Piano si sposi con le volontà di questo Governo e in modo particolare con la volontà della politica nel nostro Paese. il senatore Cervellini. Ne ha facoltà. Io credo che abbiamo il dovere di imporci di andare oltre e fare di quella tragedia l'occasione

criticare e porre l'accento sulle proposte strampalate che nei giorni scorsi abbiamo sentito fare dal Presidente del Consiglio. È forte invece il filo che le tiene, perché parla di un'assenza di cultura di fronte a questi grandi fenomeni e a queste grandi tragedie.

non ha un valore negativo in sé, ma è un messaggio che diamo, dopo aver portato anche nei mesi scorsi (e non negli anni scorsi) tutte le argomentazioni circa la negatività di un'opera di questo tipo, e non solo per le infiltrazioni della criminalità, che storicamente ha messo le sue radici in queste grandi opere. Ma io pongo una questione specifica: come si può pensare una cosa del genere? Ascoltavo con attenzione le parole del senatore a vita

Che ne è del vostro ponte davanti a una vicenda di questo tipo, al netto delle nuove tecnologie? Ma come si fa a pensare, davanti a una tragedia come quella che ha colpito ad agosto i Comuni del Lazio, dell'Abruzzo, delle Marche, di avanzare una proposta di questa natura, bloccando risorse che invece devono essere

prendevano in mano la responsabilità, la capacità, gli strumenti, le risorse, ovviamente in sintonia con gli organi dello Stato, per rimettere in piedi quella meravigliosa Regione squassata dal terremoto del Friuli. Se c'è

da aquilana ho vissuto in prima persona il drammatico sisma del 2009, le manipolazioni mediatiche e gli affarismi nazionali e locali che ha generato; e ne stiamo ancora pagando le conseguenze. Il 24 agosto la terra ha tremato ancora una volta violentemente, interessando le Province di Rieti, Ascoli Piceno e Perugia e colpendo i Comuni di Accumoli, Arquata del Tronto e Amatrice, situata a 40 chilometri dall'Aquila e a 24 chilometri da Campotosto. Dopo il risveglio da quel tragico incubo vissuto nel 2009, ci siamo trovati nuovamente a dover subire altre perdite di amici

ha provocato la tragica morte di 300 persone e ingenti danni a immobili pubblici e privati e a infrastrutture, quantificati in una prima stima del Governo in 4 miliardi di euro,

oltre a esservi la priorità di interventi legislativi per mettere in sicurezza il Paese dal rischio sismico e idrogeologico (interventi che erano stati richiesti sin dal 2009 con una proposta di legge popolare depositata e da molti di voi ben conosciuta, soprattutto dalla collega Pezzopane, e tuttavia ignorata dalle Assemblee e ignorata anche in questa legislatura), occorre procedere ad un corretto e serio riconoscimento delle aree a rischio sismico

Se si è finalmente deciso di investire sul progetto Casa Italia per la messa in sicurezza del Paese, è doveroso garantire seri criteri per la classificazione delle aree a rischio sismico del territorio nazionale. Altrimenti, se non ci sono adeguate normative tecniche, tutto viene vanificato. Il territorio dell'Aquilano, colpito da due forti eventi sismici, a Sud e a Nord, resta a oggi classificato zona 2. In quest'ottica non può bastare neppure l'obbligatorietà del fascicolo del fabbricato nelle transazioni immobiliari e relativo certificato di agibilità, ma occorre dare una corretta informazione sulla sicurezza strutturale, perché potrebbe non essere adeguato al reale rischio sismico di quel territorio e dunque necessitare di ben altri interventi per l'adeguamento sismico. In conclusione, nonostante si siano vissute tragedie analoghe a quelle di Amatrice è inspiegabile aver trascurato anche un altro aspetto negli ultimi cinquant'anni: l'importanza dell'organizzazione delle attività di soccorso, aiuto e assistenza fin dai momenti immediatamente successivi all'evento sismico. Per la salvezza di vite umane serve chi si assume la responsabilità di organizzare e dirigere gli aiuti e questo alle 3,36 del 24 agosto fino al tardo pomeriggio non è avvenuto: pomeriggio non è avvenuto: è mancato. Tutte le forze umane messe in campo per i soccorsi sono state in parte vanificate, perché nessuno ricopriva il ruolo di coordinatore delle operazioni di scavo e ricerca tra le macerie. Manca una capacità organizzativa strutturata. È vero che non possiamo prevedere con certezza quando la scossa si verificherà, ma è altrettanto vero che possiamo attribuire a livello nazionale ruoli e compiti ben definiti

Signor Presidente, è evidente che questa mattina siamo stati attirati in un piccolo inghippo procedurale: pensavamo di dover parlare del terremoto, di dover esitare degli indirizzi precisi al Governo sul futuro decreto-legge che riguarderà il terremoto (e che tarda ad arrivare rispetto alle consuetudini dei Governi

i titoli sono titoli, mentre i contenuti sono diversi da quelli che ci immaginiamo di dover affrontare. Rinvio quindi la tematica specifica del terremoto a quando vedremo arrivare effettivamente in Parlamento questo famoso decreto

tutta in sedi extraparlamentari e oggi approdata, per caso o per coincidenza di date rispetto alla presenza del collega Piano sul territorio italiano piuttosto che in altre parti del mondo, in quest'Aula del Parlamento. Abbiamo ascoltato anche alcuni interventi. Il suo intervento, molto accademico, ci ha spiegato cosa si può fare per mettere in sicurezza il nostro territorio dal punto di vista del rischio sismico. Potremmo parlare del rischio idrogeologico, come potremmo parlare anche di altre cose importanti dal punto di vista della sicurezza dei fabbricati e dei territori da ricostruire.

signor Presidente, come predisposto dal Governo Berlusconi e come poi è uscito - ora dirò per colpa di chi - dalle Aule parlamentari, leggerà che in quel decreto-legge l'articolo 11 propone l'iniziativa del controllo in tutto il territorio nazionale del rischio sismico, a partire proprio dai territori dell'Appennino centrale. Quella proposta, assieme alla proposta del successivo piano casa, fu irrimediabilmente bocciata dalla Conferenza Stato-Regioni che ne chiese e ottenne lo stralcio da quel testo. La Conferenza era all'epoca presieduta da quel Vasco Errani che oggi il Governo chiama ad essere responsabile della ricostruzione; responsabile quindi di avere differito per cinque anni - e non sappiamo poi se veramente per cinque anni perché dobbiamo ancora verificare che le proposte del collega Piano vengano accolte

che il deliberato della Conferenza Stato-Regioni stabiliva che dovevano essere le Regioni a farsi promotrici e carico di quell'iniziativa e non la Protezione civile, come indicato dall'articolo 11 del decreto Abruzzo. Non se ne fece niente perché poi le Regioni

oltre che di messa in sicurezza suggestiva attraverso i prototipi, le diagnosi dei fabbricati, tutte cose che se lei scorre, se il senatore Piano avrà la bontà di scorrere anche i disegni di legge da noi presentati all'inizio di questa legislatura... *(Brusio).* Presidente, ho ascoltato religiosamente

Non so se questo rientri nei piani di ascolto del Parlamento. Non posso certamente pretendere di essere in contraddittorio con il collega Piano. Piano. Come lui ha detto, oltre che un grande scienziato, è anche un osservatore privilegiato; dal suo studio di New York si vede l'inizio della High Line credo sia veramente privilegiato, nel senso di poter ammirare come nel mondo si evolve l'urbanistica e come si profitta anche delle cose che si dovrebbero dismettere per renderle invece assolutamente importanti e centrali rispetto ai progetti urbanistici

dei traumi per poter immaginare di fare cose utili dal punto di vista generazionale. Quindi, quando discuteremo del terremoto, dovremo discutere anche dei modelli di ricostruzione,

dove ogni anello, in base alla cultura del tempo, aggiunge qualcosa di nuovo. Vorrei fare un esempio di campanilismo siciliano. Se il principe di Biscari e il duca di Camastra non avessero immaginato, dopo il tremendo terremoto del 1693, di costruire le *new town*, noi non avremmo la Val di

abbiamo Grammichele, costruita sull'ipotesi delle città ideali di Campanella. Abbiamo un panorama culturale del mondo da dover esplorare prima di dire: ricostruiamo tutto com'era, non cambiamo un centimetro. Abbiamo veramente lavoro va fatto con un grande concorso internazionale di idee perché, così come i grandi architetti italiani sono andati nel mondo, altri grandi architetti del mondo sono venuti in Italia (Vanvitelli, per ricordarne uno). Abbiamo il dovere di dar vita ad un concorso internazionale di idee, approfittando anche del fatto le zone colpite dal terremoto dell'agosto scorso sono anche zone limitatamente cariche dal punto di vista demografico (contrariamente a quello di cinque anni fa, dove ci fu un carico demografico di persone colpite dieci volte superiore), perché questo ci può dare l'opportunità anche di esplorare modelli assolutamente nuovi, ma compatibili con il paesaggio e con la cultura italiana. Quindi la diagnosi dei fabbricati va bene ma il fascicolo del fabbricato va malissimo se viene posto a carico dei proprietari che già hanno visto negli ultimi quattro anni quintuplicare le imposizioni fiscali sugli immobili. Non vorremmo che questo fascicolo del fabbricato a carico dei proprietari degli immobili diventi un'ulteriore tassa occulta. Mentre sarebbe assolutamente importante che fosse il Governo a farsi carico dei modelli, come ci ha detto il collega Piano, dei prototipi di intervento sul patrimonio sul patrimonio immobiliare italiano. Questo lavoro va fatto sicuramente con una dimensione prospettica, ma anche con una dimensione di concretezza dal punto di vista delle delle politiche di bilancio. Ripeto, se cinque anni fa si è persa l'opportunità di iniziare a farlo, è stata colpa di quei signori che siedono sui banchi della sinistra che allora comandavano la Conferenza Stato-Regioni. Alcune cose ho potuto dirle nel tempo che mi è stato concesso per intervenire. Spero che il collega Piano voglia onorarci della sua presenza quando discuteremo del decreto-legge sul terremoto, perché con il senso della concretezza che ci ha ricordato dovremo affrontare tra poco anche l'arida l'arida argomentazione dei numeri e delle proposte; dovremo affrontare il dibattito con gli enti locali, che anche cinque anni fa

questioni che dalle esperienze del passato possono ricavare certamente elementi positivi, ma che hanno bisogno di essere urgentemente definite, e non messe ancora in attesa dopo più di un mese da quell'evento, con un decreto di serio intervento da parte del Governo. Presidente, signor sottosegretario De Vincenti, colleghi senatori, senatore Piano, abbiamo voluto con forza questa sessione di lavoro

l'urgenza di fare presto, di intervenire e di sapere, nonché la generosità e il coraggio che sono stati più forti della paura e della disperazione, e che hanno messo in salvo migliaia di persone. Era ancora buio quella mattina quando già i volontari della Protezione civile, i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine, tantissimi semplici cittadini, i sindaci, gli amministratori comunali erano in giro per i loro territori a verificare l'incolumità dei propri concittadini

per l'etica civile, l'altruismo e la determinazione dimostrati, che ancora una volta ha suscitato l'ammirazione di tutto il mondo, per la dimostrazione che abbiamo dato di essere un grande Paese, innanzitutto per il senso di comunità e di solidarietà che ci unisce. Sono stati e sono impegnati negli aiuti, in questi giorni e in quelle ore, e in quelle ore, anche tante associazioni di volontariato e, con loro, tanti ragazzi richiedenti asilo, scampati alla guerra, perché la solidarietà genera altra solidarietà: questa è una lezione importantissima. Ricordo come voi la prima notte dopo il terremoto, il dolore angosciante per le vite spezzate, per chi non c'era più, inghiottito dalle scosse e dalle macerie. In migliaia quella sera, come sappiamo, non poterono rientrare nelle loro è stato così per ogni sera: ancora adesso sono 4.454 le persone assistite e ospitate nei campi e nelle strutture allestite, nelle Marche, nel Lazio e in Umbria, grazie alla tempestività del Governo, all'impegno del presidente Renzi, del ministro Delrio, del sottosegretario De Vincenti, del commissario Errani, dei Presidenti di Regione, grazie alla loro presenza costante vicino alle popolazioni. Anche per questo la fase di emergenza sta, via via, lasciando spazio a quella della riorganizzazione e della sistemazione delle famiglie in strutture ospitali,

le persone trasferite in abitazioni provvisorie e in strutture alberghiere. Il terremoto ha colpito duramente l'entroterra, i borghi appenninici, che sono magnifici,

Se sapremo prenderci cura di noi e delle nostre case, come con grande forza e lungimiranza diceva il senatore Renzo Piano questa mattina, della qualità costruttiva e urbanistica, allora non sarà il terremoto ad allontanarci dalle città che abbiamo costruito e che sono un pezzo fondamentale dell'identità e della cultura di ognuno di noi e del nostro Paese. La prima cosa da fare è rimettere in piedi le comunità locali e permettere loro di vivere. Bisogna riattivare i servizi essenziali, gli ospedali e le scuole innanzitutto e dare sostegno alle imprese e ai lavoratori: penso a misure straordinarie per chi e ad una zona franca di *no tax area* per il rilancio delle attività produttive e per la riattivazione delle attività turistiche e culturali. Penso al sostegno alle attività

un progetto che pensi i luoghi colpiti come vivi e vitali e che veda protagonisti i sindaci, con loro le popolazioni, nelle scelte da compiere. Serviranno trasparenza, tracciabilità di ogni operazione, legalità, equità nelle scelte e rispetto dei criteri. Serviranno risorse certe del bilancio dello Stato e del bilancio europeo. Non taglieremo le nostre radici e ricostruiremo tutto com'era e dov'era. Dovremo allora investire in prevenzione del rischio sismico e idrogeologico e nella messa in sicurezza del nostro patrimonio pubblico, a partire dalle scuole, dagli ospedali, dalle case popolari,

accantonati, permettendo ai singoli cittadini di avere accesso al credito per poter utilizzare gli sgravi fiscali per la messa in sicurezza e la ristrutturazione, mettendo le centro di questo grande progetto strutturale che può dare più forza al Paese. La sfida è far rinascere i nostri borghi; lo si deve alle tante, troppe vittime sepolte nelle loro case, e dipenderà dall'impegno di ognuno di noi non far spegnere i riflettori e ad affrontare insieme un autunno e un inverno che saranno molto difficili. Il terremoto del 24 agosto è una ferita enorme e sta a noi anche saperla suturare. Il progetto Casa Italia vuole evitare che altre ferite vi siano, e oggi votiamo votiamo questa mozione con il pensiero ad Amatrice, ad Arquata, ad Accumuli, ai Monti Sibillini, alla via Salaria: luoghi amatissimi da noi marchigiani, noi laziali, noi umbri, noi abruzzesi, legati da questo pezzo di Appennino. Luoghi che sono un pezzo di noi stessi, oggi spezzati e lacerati, e che a noi tocca di nuovo ricostruire e legare insieme. che i senatori Vaccari, Marinello, Romano e Mazzoni hanno presentato l'ordine del giorno G3. Conseguentemente, sono state ritirate le mozioni nn. 620, 631 e 635. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni e sugli ordini del giorno presentati. Signor Presidente, ringrazio tutti i senatori intervenuti in questo dibattito, un dibattito importante che si sofferma a ragionare e a dare indicazioni e proposte per fronteggiare un evento drammatico, quale è stato il terremoto del 24 agosto,

Quella notte del 24 agosto la ricordiamo tutti e ricordiamo tutti il senso di angoscia nell'avvertire

già nelle prime ore di aiutare nell'azione di soccorso - hanno dato una prova straordinaria di efficienza, di efficacia di vera solidarietà. Sì, perché la solidarietà nei confronti dei cittadini italiani colpiti da quel terremoto si misura sulla capacità di

Segnalo che il Comitato operativo nazionale si è riunito

e i sindaci e le popolazioni dei paesi colpiti sanno bene che quello che sto dicendo è vero. dunque, una fase di soccorso immediato importantissima, perché il primo obiettivo era salvare vite umane. Poi, c'è stata l'assistenza alla popolazione in condizioni naturalmente di emergenza; l'immediata costituzione delle tende per ospitare quanti non potevano rientrare nelle loro case, l'assistenza sanitaria. C'è stata una mobilitazione complessiva che ha consentito di limitare i pur pesanti danni causati soprattutto, purtroppo, alle persone. L'azione per fronteggiare l'emergenza è proseguita in queste settimane. Abbiamo potuto, come ci eravamo impegnati a fare, riattivare l'attività scolastica nei tempi previsti tempi previsti e abbiamo portato sostegno e supporto agli imprenditori e ai lavoratori di quei territori. Penso, per esempio, agli allevatori, che hanno vissuto e stanno vivendo una situazione particolarmente difficile, con i quali condividiamo l'azione per consentire di gestire la situazione, di portare avanti e tutelare gli allevamenti coinvolti, ma non solo, anche l'insieme delle attività economiche. Oggi siamo impegnati nel superare la fase delle tendopoli per poter avviare la fase in cui

Questa è la fase dell'emergenza, che gestiremo fino a consentire la piena ripresa della vita quotidiana nei territori colpiti dal terremoto, e parallelamente abbiamo avviato la fase della ricostruzione nominando il Commissario straordinario per la ricostruzione che, in un rapporto molto forte con i Presidenti delle Regioni, con i sindaci e con le comunità locali ne sta delineando gli interventi e le linee portanti. Intendiamo raccogliere fino in fondo la richiesta che ci viene dai cittadini delle zone colpite: la ricostruzione dovrà avvenire negli stessi luoghi; i borghi andranno ricostruiti come erano, mantenendo la loro identità culturale e storica, naturalmente con una messa in sicurezza antisismica che risponda agli*standard* che le tecnologie attuali consentono finalmente di realizzare. Il contributo che è venuto dal dibattito di questa Assemblea stamattina sarà prezioso per l'elaborazione, che è già in corso, delle norme che intendiamo varare con un prossimo ravvicinato provvedimento, che faranno da cornice normativa a tutta l'azione di ricostruzione nelle aree terremotate. sostegno alla ricostruzione delle prime case, ma anche delle seconde case, perché in quei territori le seconde case significano attività economiche

Il decreto-legge tratterà la ricostruzione delle aree terremotate. E poi c'è una strategia più generale che abbiamo chiamato Casa Italia:

abbiamo dedicato - per esempio - per la banda ultralarga, per il dissesto idrogeologico, per l'edilizia scolastica o a quelle previste nel *masterplan* per il Mezzogiorno. Quelle risorse già ci sono. La legge di stabilità le sistematizzerà e ne aggiungerà altre. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno cominciato a lavorare sul progetto Casa Italia e primo fra tutti il senatore Renzo Piano, il quale nel suo intervento di oggi ci ha confermato una disponibilità preziosa per l'elaborazione delle linee portanti della mappatura e messa in sicurezza del nostro Paese, quel rammendo di cui ha parlato che è fondamentale perché - come il senatore ci diceva prima - dobbiamo essere consapevoli di quali bellezze il nostro Paese contenga e di che patrimonio sia l'Italia per l'umanità Voglio ringraziare anche il professor Giovanni Azzone, rettore del Politecnico di Milano, che ha accettato di guidare l'unità di missione Casa Italia e che sta raccogliendo i contributi che, a partire da quello del senatore Piano, stanno arrivando dagli istituti di ricerca, dalle forze economiche e sociali e da tutte le istituzioni. È in atto un lavoro corale, condiviso, che è quello che serve per avviare finalmente la nuova strategia per il nostro Paese.

che oggi vede insieme il Partito Democratico con NCD e anche AL-A. Il Governo, che in questo momento è rappresentato solo dal sottosegretario De Vincenti (essendo il Presidente del Consiglio dei ministri dipartito appena terminato l'intervento del senatore Renzo

Ovvero, si dichiara contrario all'istituzione di una zona economica speciale, come la Lega richiede, affinché in quelle zone possa ricostruirsi un tessuto economico che garantisca alla gente di poter vivere e ricostruire le attività produttive. si ritiene contrario alla nostra proposta di chiedere il rinvio del pagamento degli oneri previdenziali, di chiedere che non vengano lasciati in capo a chi è oggi terremotato oneri che maturano che maturano anche interessi sui mutui e altri oneri che non sono in grado di pagare. Questo oggi noi chiediamo qui dentro. Io avrei preferito - e sarebbe stato molto più coerente da parte del Governo la richiesta a tutti i Gruppi di opposizione di partecipare alla stesura di un documento unitario: proposta che non abbiamo sentito sottoporre. E ciò dimostra che l'obiettivo vostro qui dentro oggi, ancora una volta, non era trovare l'unità del Paese per dare una risposta forte e seria rispetto al terremoto e alla futura prevenzione. Il vostro obiettivo - come avete ben declinato era solo realizzare uno *spot* preelettorale per potere convincere magari qualcuno, truffaldinamente, sulle capacità del Governo. del Governo. Altrimenti, non riusciamo a capire la presenza istantanea di Renzi, a parte per prendere il cappuccino, ai fini di ascoltare solo l'intervento del senatore Piano, come se tutti gli altri qui dentro fossero degli sciocchi e non meritassero l'attenzione da parte del Governo.

consentendo a chi oggi è ancora nelle tende in attesa che gli venga data una struttura fissa di rimanere accanto ai propri allevamenti e alle proprie case. Chiediamo una cosa banale, semplice: le pene previste per lo sciacallaggio e per gli altri delitti infami che vengono compiuti nelle aree colpite dal terremoto devono essere elevate. Questo è un ulteriore segno di inciviltà. E su questo si può dire di no?

Cosa è il ponte sullo Stretto se non uno *spot* preelettorale? Usate quei soldi per dare sicurezza a tutti gli altri Comuni della fascia appenninica che sono nelle stesse condizioni di Amatrice. Allora farete una cosa seria, altrimenti è solo uno *spot* elettorale.

svolgere una dichiarazione di voto, perché pensavo che su un tema come quello del terremoto ci sarebbe stata, nel dibattito in Aula e da parte del Governo innanzitutto, tutta la disponibilità a condividere alcune delle buone

che tutti i Gruppi hanno proposto mozioni con l'intento e con l'obiettivo di portare sollievo a quelle popolazioni e anche di affrontare il tema più ampio del dissesto del nostro territorio, della sua fragilità, della sua delicatezza nel caso specifico di Amatrice,

Il Governo è contrario agli ecobonus e agli incentivi fiscali? No. Eppure, in tutte le mozioni c'è questo e anche molto altro. Penso che le parole del collega Candiani abbiamo messo in evidenza solo una parte del problema, parte del problema, che è un po' più ampio. È possibile che persino il terremoto debba essere considerato l'occasione di una divisione

comunicazione che, anche attraverso l'utilizzo del povero senatore Renzo Piano, viene strumentalizzata dal Governo per potere illudere che questa sia la volta buona e che si può trovare una soluzione diversa rispetto a quelle del passato. ho un timore, visto il copione che si va ripetendo e vista l'indisponibilità davvero strana da parte di un Governo che non vuole raccogliere attorno a sé tutte le tutte le forze politiche per poter avere il sostegno e compiere uno sforzo ulteriore e magari migliore di quello di Governi precedenti per dare risposte. E penso, penso, allora, che le parole del collega Candiani siano un po' forti, ma diano esattamente il senso di quanto è andato in scena in Aula questa mattina. Mi dispiace che il sottosegretario De Vincenti non colga l'opportunità di avere il sostegno di larga, larghissima parte di questo ramo del Parlamento

dagli effetti di un'azione di Governo che non so se si realizzerà, ma di certo parte sola, isolata nella sua stretta o larga maggioranza, a seconda delle sedute e delle giornate. Si tratta di una maggioranza che, alla fine,

colleghi, ritengo anzitutto che sia un fatto molto positivo che, appena calata la polvere delle case crollate nell'ultimo terremoto, il problema della sicurezza antisismica e della lotta al dissesto idrogeologico non sia stato rapidamente derubricato a tema di ordinaria amministrazione, come più volte è avvenuto Uno strumento da cui partire esiste già ed è il Fondo per la prevenzione, approvato all'indomani del terribile terremoto dell'Aquila del 2009.

delle abitazioni private sono un'assoluta rarità: c'è, infatti, l'obbligo solo per le nuove costruzioni o per le ristrutturazioni importanti. Tuttavia, se si guarda a quanto ha speso lo Stato italiano negli ultimi per le ricostruzioni dopo i terremoti, si scopre che un grande piano di consolidamento antisismico avrebbe fatto risparmiare. Quindi, lo Stato ha speso molto, ma male, agendo sempre sull'onda delle emergenze e mai in modo strutturale per un'adeguata prevenzione. davvero il momento di cambiare registro, e non solo con il progetto Casa Italia, che avrà inevitabilmente un orizzonte di lunga durata, ma con la stessa legge di stabilità che approveremo a dicembre. i Governi che si sono succeduti hanno stanziato nel Fondo per la prevenzione del rischio sismico una somma complessiva inferiore al miliardo di euro, mentre nello stesso periodo il valore degli importi detraibili per la sola riqualificazione energetica - ossia l'ecobonus - ha superato abbondantemente i 12 miliardi

una sostanziosa detassazione degli investimenti privati nel consolidamento antisismico andrebbe probabilmente nella giusta direzione. Allo stesso modo, sarebbe opportuno istituire un'assicurazione obbligatoria sulla casa, totalmente detraibile dalle tasse, che copra, tra gli altri, anche i rischi derivanti dalle calamità

prevedendo a fianco dell'indispensabile intervento pubblico l'entrata in scena di soggetti terzi come le compagnie assicurative - magari coordinate da un'autorità pubblica - le quali, per tutelare i propri interessi, spingerebbero gli assicurati a comportamenti responsabili tesi a contenere gli effetti dei disastri della natura.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il terremoto del 24 agosto scorso, drammatico per intensità, intensità, tragico e doloroso per centinaia di persone, ha segnato una continuità prevedibile con la riconosciuta sismicità di una vasta area del territorio nazionale. Tuttavia, ha segnato anche la manifesta solidarietà di tantissimi che, a vario titolo, hanno partecipato e sono intervenuti immediatamente. L'impegno alla ricostruzione richiederà evidentemente dei tempi. L'attesa e la fiducia riposta, sulla base degli impegni assunti ai più alti livelli istituzionali, non saranno certamente disattese. Ma la ricostruzione del tessuto urbanistico non può ritenersi congrua se non si fonda su una rinnovata coesione sociale una robusta visione di comunità, dove il capitale sociale è protagonista e interprete prima, destinatario da subito. Ritengo che questa sia la sfida che il terremoto ci pone. Casa Italia è un progetto ampio per obiettivi e provvedimenti che consentano ricostruzione, adeguamento antisismico, investimenti sul dissesto idrogeologico e, soprattutto, ragionevole prevenzione a partire dagli edifici pubblici. Per alcuni questo progetto è utopistico, irrealizzabile, intriso e connotato di buio disincanto. Eppure, ritengo fermamente che sia fattibile, seppur in tempi che non possono essere certo brevi. Ma ritengo ancor più che Casa Italia è tale se sa essere casa solidale, ovvero comunitaria partecipazione, appunto condivisa, in responsabilità. Una ricostruzione che non sia solo funzionale sotto il profilo ingegneristico e architettonico può e deve basarsi sulla sostanziale ricostruzione di un tessuto sociale fatto di storie, di umanità, di memorie e speranze, aspettative e investimenti. È storia di persone, che insieme e non da sole possono costruire un futuro degno di quelle terre, della nostra Italia. Casa Italia, quindi, è un simbolo, può rappresentare un simbolo ed è la rappresentazione di una fiducia, appunto comunitaria, dove ognuno sia partecipe, facitore e quindi attore in sussidiarietà e responsabilità.

saranno espressi, da parte del Gruppo Per le Autonomie, consenso e favore. Mi riferisco ai paradigmi della qualità, della democrazia, della trasparenza, della legalità e dell'equità: il paradigma della qualità massima e dell'efficienza degli interventi, con il massimo rispetto possibile dell'identità dei luoghi e degli edifici; democrazia attraverso una responsabilizzazione delle comunità locali e di tutti i livelli istituzionali presenti; trasparenza per mezzo di piattaforme informatiche per la gestione di tutte le risorse e la rendicontazione puntuale e continua degli interventi; legalità attraverso la creazione di meccanismi di selezione e continuo controllo puntuale delle imprese incaricate dei lavori; infine, non ultima, equità, ovvero corresponsione del dovuto ai cittadini, alle imprese e agli enti delle comunità colpite, in un principio quindi che sia rispettoso di tutti e ci dia la possibilità di una ricostruzione

che quella odierna potesse essere un'occasione di confronto serio e nel merito. Abbiamo apprezzato l'intervento del senatore Piano, che ci ha ricordato quanto sarebbe importante nel nostro Paese investire non solo genericamente nella messa in sicurezza, ma anche nella custodia delle sue bellezze paesaggistiche e culturali. Invece, purtroppo, signor Presidente, devo prendere atto che, ancora una volta, sono stata disillusa. Lei mi dirà che sono molto ingenua. Io non sono tanto ingenua, ma cerco sempre di avere una sorta di ottimismo della volontà. Non mi sfuggiva che oggi si sarebbe tentato di mettere in onda una sceneggiata, con la comparsa del Presidente del Consiglio e del grande architetto, tutto apparecchiato per una comunicazione esterna di propaganda.

a dir poco ‑ di utilizzare la questione del terremoto per fare altre operazioni e non per dare risposte precise alle persone

cambiare completamente, fare un cronoprogramma, una pianificazione seria di tutto quanto è necessario fare.

in quest'Aula in cui tutto viene finalizzato esclusivamente alla propaganda? Guardate che così non è assolutamente possibile. Ma state attenti, perché i cittadini a questo punto cominceranno a stufarsi veramente. Anche oggi abbiamo svolto un dibattito che non era per i terremotati ed era finalizzato non a intervenire

una ricostruzione che abbiamo chiesto debba essere rispettosa dell'ambiente, del linguaggio architettonico e, in un certo qual modo, eviti le libere interpretazioni sul tema che tante volte hanno caratterizzato altre aree e hanno portato alla costruzione delle cosiddette cattedrali nel deserto;

Governo, nella ricostruzione e anche nella grande idea di Casa Italia, che non è soltanto la messa in sicurezza - come dicevo poc'anzi nel mio intervento precedente - dell'edilizia pubblica e privata, ma anche una sorta di approccio sistemico a tutte le problematiche del territorio. territorio. Il coordinamento deve essere prevalentemente politico più che operativo, proprio per evitare la duplicazione di una serie di organismi che molto spesso non hanno dato o non danno buona prova di sé. Penso anche alla struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, sul quale personalmente avanzo una serie di dubbi. In ultimo, vi è il coinvolgimento, Sottosegretario, degli ordini professionali, sicuramente organi ausiliari dello Stato che - a mio avviso - vanno quindi coinvolti a pieno titolo. Infine, a proposito di prevenzione, bisogna attivare il sistema dei controlli e delle verifiche. Alcuni decenni addietro, quando si doveva collaudare un'opera in cemento armato, sia pubblica che privata, esisteva un albo dei collaudatori gestito direttamente dalle prefetture e con criteri di assoluta terzietà.

possano innescarsi conflitti di interesse che spesso sono la causa o comunque sono alla base di alcuni disastri che abbiamo registrato anche nell'ultima disgrazia. Detto questo, confermo il voto favorevole di Area Popolare. Dopodiché sarà compito della politica trovare delle ragioni forti che - a mio avviso - su tematiche di questo genere non possono assolutamente essere né divisive, né demagogiche, né populistiche.

voi state facendo riferimento a qualcosa che ancora non esiste, il progetto Casa Italia (che somiglia tanto al "progetto casa" di qualcun'altro), e demandate il reperimento di risorse a quanto verrà in esso scritto.

I soldi allora ci sono per questo e non per altro. Sento poi parlare di tutta una serie di impegni che riguardano la prevenzione, le *white list*, la democrazia nella scelta delle ricostruzioni. Ma è dal 1980 e dal terremoto dell'Irpinia che sento dire esattamente le stesse cose. Alcuni di voi hanno avuto incarichi di Governo, siete stati in Parlamento e dite ancora le stesse cose. Perché non le avete fatte? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Siamo ancora al punto in cui bisogna impegnare il Governo a fare una cosa a cui doveva arrivare da solo. Ma che impegno sarebbe questo? Di cosa stiamo parlando? Giusto per la questione delle risorse, a chi pensa che sia una buona idea fare il ponte sullo Stretto di Messina, voglio ricordare il *tunnel* sotto la Manica e il suo rientro economico, che non c'è mai stato. Vogliamo fare un ponte da 10 miliardi solo per avere l'appoggio di Salini Impregilo alla revisione costituzionale in cambio di un debito perpetuo per lo Stato? Vogliamo veramente fare questo? Complimenti! E poi mettete assieme la riqualificazione sismica con la riqualificazione energetica, ma cosa? Prima la riqualificazione sismica. Attenzione: voi continuate a fare riferimento alle mappe della sismicità che sono strumenti probabilistici, misurano la probabilità che un terremoto superi una certa intensità in un arco temporale di cinquanta anni e non vedono il picco. Per questo a Fukushima, costruita con tutti tutti i crismi, è successo quello che è successo. Milano si trova in zona 3, una zona quindi di sismicità bassa. Peccato che nel bresciano c'è stato un terremoto di magnitudo 5.5, tanto tempo fa, ma c'è stato. Qual è l'orizzonte temporale di questi interventi? Allora ha ragione Delrio

i terrapieni sottostanti all'ingresso del ponte, ho fatto un ponte antisismico che non può più essere usato perché non ci si può arrivare. E allora di cosa stiamo parlando? Questi ragionamenti sono roba da scuola elementare. Andiamo avanti. la flessibilità all'Unione europea, andiamo ancora a chiedere soldi all'Unione europea? Ma un bel "vaffa" all'Unione europea, no? Dico che è il momento di dirlo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La flessibilità l'avete chiesta per gli 80 euro, per le clausole di salvaguardia e anche per il *jobs act*, per cercare di racimolare consenso. Per questa roba, non chiedo la flessibilità, ma prendo quello che devo prendere. Se non gli sta bene, me ne frego.

dà più di quello che prende. Tu mi fai una multa di 300 milioni, ti do 300 milioni in meno, cosa mi fai? Mi invadi? Fai una guerra commerciale e me che sono il tuo *partner* importatore che compera da te? Siamo noi che li teniamo per le palle, non loro. E facciamo il contrario? *(M5S)*. Concludo. Noi chiedevamo e chiediamo una cosa molto semplice: soldi sul tavolo chiari già dalla legge di stabilità, un fondo rotativo perpetuo. Il patrimonio immobiliare che avevamo è completamente da risistemare, infrastrutture comprese. Qualcuno ha detto, e non ha sbagliato del tutto, che questo tipo di investimenti genera un volano positivo per l'economia; ci sono tutti i moltiplicatori che lo dicono, però vediamoli, questi soldi. Perché dobbiamo rimandare ad un fantomatico progetto Casa Italia che è un contenitore vuoto? Questo è il momento di chiedere loro di mettere i soldi sul tavolo, e non di aspettare un'altra volta e Mi sono stancato di vedere questa cosa piana, voglio vedere i soldi, mucchi di soldi. Invece del ponte, i soldi li voglio vedere qui. Signor Presidente, onorevoli senatori, membri del Governo, siamo qui a discutere di fronte all'ennesima tragedia

noi non intendiamo strumentalizzare in alcun modo tragedie come queste. Ricordiamo la vergognosa azione portata avanti dalle forze dell'opposizione rispetto al quarto Governo Berlusconi, che è stato l'unico ad avere destinato fondi a favore dei territori colpiti dal terremoto in Abruzzo, e la fase di ricostruzione gestita dai successivi Governi è stata lunga, travagliata e ancora non completamente portata a compimento. Di fronte a situazioni come queste, la prima cosa da fare è una ricostruzione rapida ed efficace dei territori danneggiati. bisogna trovare delle soluzioni per ridurre le calamità naturali che in questo Paese avvengono in maniera troppo frequente. i tagli operati dal Governo agli enti locali oramai impediscono quel minimo di manutenzione che serve nei territori, perché non si puliscono più i canali, non si mettono a regime i fiumi alla fine, ad ogni acquazzone un po' più violento rispetto al normale, ci troviamo di fronte a delle tragedie umane. Dicevo che la prima cosa che dovrebbe fare il Governo è quantificare i danni, perché ho sentito cifre di 3 o 4 miliardi, mentre io posso dire, visto che abito nel territorio delle Marche, che i danni questa volta sono più ingenti del terremoto che ha colpito l'Umbria e le Marche

bisogna fare una programmazione pluriennale delle risorse necessarie per riparare i danni accaduti.

urgenti per favorire l'immediata ricostruzione e la ripresa della normale attività del tessuto economico e sociale delle zone colpite dal sisma. L'altra cosa che credo sia necessaria - ho visto che il decreto non è uscito e penso che stia per uscire - è semplificare le procedure, tutte le procedure, perché è un problema anche rimuovere i detriti derivati dal sisma: i cittadini che vogliono intervenire nella loro casa non sanno dove portare i detriti, perché questo è già un problema. Inoltre, chi ha costruito un alloggio di fortuna perché ha avuto regalata una casa di legno, oggi si trova ad avere realizzato un abuso edilizio, Poi credo che una riflessione vada fatta sull'edilizia scolastica. Noi continuiamo ad imbiancare gli edifici scolastici costruiti con l'utilizzo di materiali poveri ma anche se li imbianchiamo non sono in grado di resistere alla furia degli eventi sismici. Bisognerà pensare a ricostruire questi immobili, che non debbono essere adeguati alle norme antisismiche, ma ricostruiti di nuovo.

è chiamato a svolgere una delle sue funzioni primarie, spesso sacrificata al lavoro legislativo quotidiano, che è quella dell'indirizzo politico, che i rappresentanti del popolo hanno il diritto e il dovere di dare al Governo. Non possiamo non ribadire, accanto al ringraziamento ai soccorritori, lo sgomento, il dolore e il cordoglio per quest'ultima tragedia, che si aggiunge a quelle che hanno accompagnato l'evolversi della nostra storia nazionale, entrando - come si suol dire - nel nostro DNA, quello di un popolo che sa sorridere, che sa far sorridere, ma che porta dentro un dolore non sopito, una malinconia latente, frutto di una storia lunga di dolore, di fatica, di lotta per le conquiste e per la liberazione dal bisogno, dalle ingiustizie e dalle calamità naturali. Abbiamo ricordato tutti, in questo mese, le tragedie degli ultimi cinquant'anni, dall'alluvione del Polesine fino al terremoto del 24 agosto, dimenticare i 30.000 morti del terremoto della Marsica immortalati da Ignazio Silone, e i 100.000 che sette anni prima di quel tragico 1915, che segnò l'avvio dell'inutile strage della Prima guerra mondiale, colpirono Messina e la Calabria in quello che forse è il più grande terremoto della storia dell'umanità. Questa memoria non ci deve servire per piangere e per compiangerci, ma per capire che fare e decidere il da farsi. Questo è lo spirito e lo scopo dell'ordine del giorno G3, che stiamo per approvare e che i colleghi Vaccari, Marinello, Lucio Romano e Mazzoni hanno presentato. Il Gruppo del PD lo voterà convintamente, voterà convintamente, insieme agli impegni in esso contenuti, perché quarant'anni dopo il terremoto del Friuli, che fece capire la necessità di avere un adeguato sistema di protezione civile per affrontare le emergenze, fin dal livello comunale, occorre oggi avere una prospettiva più ampia, sintetizzata sintetizzata con le parole progetto Casa Italia i cui obiettivi sono stati illustrati anche dal senatore Piano. Come ricordava il presidente Zanda nel suo intervento del 13 settembre, nessun Governo che si è alternato in questi settant'anni di Repubblica ha avuto la lungimiranza di avviare un programma di lungo periodo per mettere in sicurezza le parti più fragili del nostro Paese, che in pochi decenni ha visto aumentare di 20 milioni la sua popolazione, in un territorio di soli 300.000 chilometri quadrati, in buona parte rappresentato da montagne, e che in soli venti anni, tra il 1950 e il 1970, è passato dall'essere un'economia sostanzialmente agricola, con qualche area industrializzata, a diventare la settima potenza industriale del mondo. Questo sviluppo, che pure ha generato il benessere di cui tutti abbiamo goduto, ha prodotto distorsioni che vanno corrette con il rafforzamento sì degli strumenti emergenziali, ma soprattutto con interventi che rimarginino le ferite di un'urbanizzazione disordinata e di scarsa qualità, di un dissesto idrogeologico dovuto anche allo spopolamento della montagna, di edificazioni non rispondenti a criteri di sicurezza. Occorre una svolta, e accanto a una normativa quadro omogenea in tutt'Italia, quale quella contenuta nel progetto di legge alla Camera dell'onorevole Chiara Braga e di altri, che mira a rafforzare un quadro omogeneo e un sistema di protezione civile, accanto al potenziamento del fondo per la prevenzione del rischio sismico, accanto alla delega al Governo per il riordino del Sistema nazionale di protezione civile, ben venga un progetto Casa Italia, che chiama tutti, maggioranza e opposizione, a volgere lo sguardo sul futuro, a mettere in campo volontà e risorse non per catturare consenso oggi - come qualcuno ha paventato - ma per restituire alle nostre comunità, in un periodo non breve, intergenerazionale, un patrimonio edilizio e un assetto urbanistico delle città che sia in grado di reggere la sfida che madre natura ogni tanto lancia all'uomo e quelle dello sviluppo che noi stessi democraticamente ci diamo. Un grande progetto che riguarda l'urbanistica, l'edilizia, il risparmio energetico, che prevede forti strumenti locali di gestione degli interventi e forti poteri di controllo centrale; che dovrebbe creare un Paese che non vuole restare indietro e che vuole valorizzare le autonomie locali, essendo unito, e che si ponga altresì lo scopo di indirizzare verso beni, che, pur privati, hanno un intrinseco valore pubblico: i consumi della gente. La politica deve saper rispondere alla domanda di futuro che le popolazioni colpite da queste tragedie le rivolgono, che ci rivolgono. Dobbiamo far capire che abbiamo capito. del giorno può aprire una fase nuova, cui ci auguriamo - proprio per le prospettive che apre di lungo periodo - voglia concorrere l'intero Parlamento, maggioranza e opposizione. Per questo il Gruppo del PD vota convintamente questi obiettivi, e si augura che intorno a questa volontà ci sia un largo consenso di tutte le forze qui rappresentate. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni. Dopo la votazione delle mozioni,

Presidente, le pongo una riflessione. Per stessa ammissione del Governo, ci sono parti coincidenti. La votazione per

Sulla mozione c'è la possibilità di votare per parti separate se c'è una richiesta e se l'Assemblea è d'accordo sul voto per parti separate. Altrimenti non possiamo che andare avanti con la votazione. Metto ai voti la richiesta

a considerare e a guardare esattamente cosa abbiamo votato e bocciato precedentemente. Passiamo dal punto di vista procedurale lei poco fa ha posto in votazione le mozioni precisando che sarebbero state votate nell'ordine di presentazione, salvo le parti che fossero risultate precluse dalle votazioni precedenti. Lo ha detto lei e lo possiamo verificare tra poco sul Resoconto stenografico. Adesso lei si rimangia quello che ha detto.

il voto a "pacchetto completo", adesso noi non possiamo andare a votare di nuovo le parti delle mozioni, come lei ha detto, che sono già comprese. Sono d'accordo, ma questo giochino di respingere le proposte sensate del Movimento 5 Stelle per ripresentarle in maniera surrettizia deve finire! Dovete prendervi la responsabilità di ciò che fate negando le cose di buonsenso. persone corrette di fronte ai cittadini.

il voto elettronico,

un uomo che ha dedicato tutta la sua esistenza alla politica. In un momento in cui la politica è in crisi perché non c'è più rapporto

dalla Democrazia cristiana ad oggi, ma soprattutto è stato un amico di tanti di noi che hanno condiviso la sua passione. Per questo credo che ricordare Michele Forte rappresenti un atto di grande consapevolezza istituzionale e anche un dovere personale e morale.

che era una politico di razza, che faceva la politica sul territorio. Al di là delle differenti appartenenze politiche, con Michele Forte ci siamo sempre confrontati,

La sede Almaviva di Palermo, che vede due siti operativi dal 2001, gestisce i servizi di assistenza telefonica per clienti quali TIM, Vodafone, Wind e molti altri, quali Alitalia, Trenitalia ed ENI, occupando circa 5.000 addetti. Pertanto, *in primis* le forti preoccupazioni per il futuro dei lavoratori coinvolti riguardavano, per l'appunto, proprio la salvaguardia dei posti di lavoro. La cosiddetta vertenza Almaviva rappresentava evidentemente un'emergenza sociale, considerato inoltre come la mancanza di una politica industriale condanni la regione Sicilia

sulle gare al ribasso al di sotto del costo del lavoro e su tutte quelle distorsioni o anomalie che soffocano le aziende del settore le quali, a loro volta, fanno ricadere le conseguenze sui lavoratori alterando, al contempo, le condizioni per una corretta concorrenza. Dalla stampa si apprende come, ad oggi, non siano ancora pervenute quelle risposte tanto attese dall'accordo risalente all'agosto 2013, tanto da portare le segreterie nazionali di tutti i sindacati,

Il punto è che Almaviva ha già inviato le raccomandate ai suoi dipendenti, per un trasferimento che avverrà il 24 ottobre, cioè quattro giorni dopo. Esortiamo che l'incontro avvenga un po' prima, in modo da trovare una soluzione. Tale richiesta origina dalla decisione di Almaviva, comunicata ai sindacati di cui sopra, di procedere ai primi trasferimenti unilaterali dei lavoratori impiegati nella commessa ENEL dalla sede di Palermo. Come ho già detto, le lettere sono arrivate e il 24 ottobre e alcuni di loro dovranno dirigersi verso la nuova sede che in provincia di Cosenza, cioè in Calabria, comunque lontano dalla sede palermitana e sicuramente per i lavoratori non è un posto agevole. Il trasferimento collettivo dei 396 dipendenti di Almaviva Contact di Palermo impegnati nella commessa ENEL rischia di essere un licenziamento mascherato, che sconfessa l'accordo del 30 maggio per il mantenimento dei livelli occupazionali dell'azienda. Il trasferimento voluto dall'azienda mal si concilia infatti con le posizioni dei lavoratori coinvolti: lavorare a Palermo o in Calabria per

una buona sintesi per mantenere entrambe le posizioni.

della Lega Nord sono diverse da quelle del Governo, che ha deciso di accogliere un fiume di persone che cercano fortuna nel nostro Paese, imponendo l'inserimento in tutto il territorio nazionale di centri di accoglienza con metodi abbastanza senza coinvolgere i sindaci e senza dare informazioni alle comunità. Esistono quindi delle differenze sostanziali, tuttavia chiediamo al Governo che nella che nella gestione di questo fenomeno, che noi non condividiamo su tutta la linea, venga utilizzato almeno il buon senso. È inaccettabile che, a fronte degli afflussi ormai inarrestabili dal Nord Africa, il Governo non impedisca che in un dato territorio ci siano concentrazioni eccessive di centri di accoglienza e di profughi.

che attualmente governa le sorti della comunità di Abano, in accordo con il prefetto di Padova, ha invece cancellato, intendendo realizzare in questa caserma dismessa il predetto *hub*. Ricordo che nel territorio vicino, cioè a Cona e a Bagnoli di Sopra, due piccoli Comuni delle province di Venezia e di Padova, ci sono degli *hub* che ospitano fino a 2.000 profughi. È quindi evidente a tutti che, a fronte di una politica scellerata, non c'è limite al peggio da parte dei prefetti e del ministro Alfano, che non colgono almeno la necessità di non creare questi insediamenti così affollati e vicini, tanto da suscitare la rabbia della gente. Non è più una protesta, ma una vera rabbia. Ci sono state manifestazioni da parte di migliaia di cittadini in quei territori c'è un ricorso contro l'agire del commissario prefettizio. C'è ormai un'insofferenza che rischia ormai di diventare esplosiva. Siccome non vogliamo che si arrivi a questa situazione, chiediamo un impegno formale - e non parole generiche, come quelle espresse ieri il *question time* alla Camera dal ministro Alfano - a che quell'*hub* ad Abano Terme non verrà utilizzato, che si ridurrà la concentrazione di profughi nel territorio dei Comuni padovani che ho citato e che ci sarà maggiore intelligenza e attenzione da parte del Ministero dell'interno nell'affrontare questa vera e propria emergenza. Non ci siamo, non ci accontentiamo più delle parole, oltre a tutto generiche, del ministro Alfano. Vogliamo dei fatti concreti. Diciamo no all'*hub* di Abano Terme. *(Applausi della

Il Comune si sveglia ora e cerca di fare il paladino di Francia, dicendo che bisogna trovare una soluzione, mentre il MISE dichiara di voler supportare ogni percorso che possa portare a una soluzione.

pochi mesi fa ha addirittura dichiarato che ha investito un miliardo di euro in progetti destinati a rivalutare il *made in Italy*. Al MISE è stata proposta anche la possibilità di coinvolgere altre multinazionali del settore.

Dopo cosa faranno? Vogliamo dare un'altra possibilità a queste persone, che non sia quella di avvicinarsi sempre più all'orlo del baratro? Vogliamo trovare delle soluzioni fattibili? Concludo ricordando che ho chiesto lo svolgimento di un'audizione dei lavoratori in Commissione lavoro sin dal 13 maggio 2015. Vogliamo dare voce a questi lavoratori? Vogliamo trovare delle soluzioni?

di cui si parla nella mozione, con un rischio veramente grave ed importante per il settore. Questa assenza di risposte ci preoccupa molto.